gli onorevoli interroganti pongono con l'atto ispettivo l'attenzione sulla tematica della sicurezza correlata alla svolgimento di pubbliche manifestazioni ed eventi di pubblico spettacolo e sulle ripercussioni che, a seguito dell'aumento dei recenti vincoli istituiti in materia, potrebbero determinarsi sull'organizzazione di eventi o manifestazioni di più ridotta portata e a impatto esclusivamente locale. Al riguardo, informo che la questione ha formato oggetto di una recentissima rivisitazione dei criteri contenuti nelle precedenti circolari dello scorso anno, attraverso l'emanazione da parte del Ministero dell'interno della direttiva del 18 luglio scorso, indirizzata ai prefetti, con cui sono stati elaborati nuovi modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Con la nuova direttiva si è inteso ricomporre in un quadro unitario le precedenti linee di indirizzo, al fine di contemperare, da un lato, le esigenze di garanzia di adeguati *standard* di sicurezza e incolumità dei partecipanti, dall'altro, il rispetto delle tradizioni storico-culturali e del patrimonio economico-sociale delle collettività locali, riconoscendo un ruolo Le nuove indicazioni operative intendono, infatti, assicurare un approccio flessibile alla gestione del rischio, parametrando le misure di sicurezza in relazione alla "vulnerabilità" legate a ciascun evento, con l'obiettivo di rendere le prescrizioni maggiormente conformi alle peculiarità del territorio, superando in tal modo le criticità applicative delle precedenti direttive. La nuova direttiva del 18 luglio 2018 si muove, quindi, all'insegna della flessibilità. Fermo restando le ipotesi in cui è il sindaco a rilasciare il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento dell'evento, nel documento si stabilisce, infatti, che sono i sindaci o i presidenti delle commissioni di vigilanza a dover informare le prefetture circa le peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti. Contrariamente all'impostazione che caratterizzava la precedente disciplina ministeriale, oggi sostituita, aumenta, pertanto, la discrezionalità dei sindaci nella valutazione delle potenziali vulnerabilità connesse a ciascun evento. Solo a seguito, infatti, di tale segnalazione da parte del sindaco o del presidente della Commissione di vigilanza ed acquisita la documentazione prodotta dall'organizzatore, toccherà alle prefetture - qualora ne constatino l'effettiva esigenza - sottoporre l'argomento all'esame del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato alla partecipazione del comandante provinciale dei Vigili del fuoco, per analizzare in tale sede i dispositivi di *security* e quelli di *safety*, eventualmente modificando o implementando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti necessario in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza. Peraltro, a conferma della intervenuta esigenza di non compromettere lo svolgimento di eventi che nella vita di alcune comunità rappresentano fattore dì identità e di attrattività anche economica del territorio, faccio, infine, notare che nella nuova direttiva del Ministero i prefetti sono stati incaricati di svolgere per la circostanza con il coinvolgimento delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e delle altre istituzioni e realtà associative interessate - ogni più prudente valutazione, allo scopo di modulare e calibrare adeguatamente le prescrizioni in materia, per renderle in tal modo più rispondenti alle peculiarità del territorio e delle manifestazioni programmate in sede locale.

dice, l'impegno, la gestione, la decisione dei criteri sostanzialmente ai sindaci. Lei sa, signor Sottosegretario, che i sindaci spesso sono coinvolti e sono chiamati a una responsabilità più grande di quella che spetta loro. La soluzione adottata mi sembra, ancora una volta, una via di fuga per non affrontare seriamente il problema, per evitare di emanare una direttiva che offrisse criteri tali da dare sicurezza e certezza sia al mondo del terzo settore, del volontariato e delle *pro loco*, sia, soprattutto, ai sindaci che, ancora una volta, sono chiamati a una responsabilità senza avere gli strumenti e la possibilità di agire con serenità. Spesso i sindaci si assumono tante responsabilità e sono chiamati

di agire con una direttiva che dia un po' più di certezza ai sindaci e consenta finalmente al mondo del volontariato, delle *pro loco* e delle parrocchie di poter organizzare gli eventi senza troppe complicazioni, ma con alcuni indicatori certi e chiari.

i gruppi criminali nigeriani operanti in Italia sono caratterizzati da frammentazioni etnico-tribali, filiazioni di una vasta struttura criminale costituita da poche famiglie, la cui crescita è stata sostenuta dallo strategico supporto fornito da una ramificata rete di omologhi *clan* presenti sia in Nigeria che in altri Paesi europei ed extraeuropei. La struttura di tali gruppi presenta un vertice con uno o due capi di nazionalità nigeriana, che gestiscono a livello internazionale l'attività e i rapporti con altri gruppi. La base, invece, non ha una precisa connotazione etnica. Detti sodalizi, che mantengono una sostanziale autonomia nei rapporti con la criminalità organizzata italiana, sono dotati di una rete nazionale di referenti a capo di cellule di apparente connotazione folkloristica, dietro le quali si celano agguerrite associazioni criminali che, con modalità di intimidazione, controllo e violenza fisica gestiscono le attività illecite. Recenti attività investigative, condotte dalle Forze di polizia, hanno confermato come le consorterie in parola abbiano assunto, in taluni casi, la conformazione di vere e proprie associazioni per delinquere, utilizzando *modus operandi* tipici delle mafie autoctone. Particolare attenzione, da parte degli investigatori, è riservata ai gruppi degli Eiye e dei Black Axe, nonché alle componenti nate da loro scissioni, riconducibili ai Secret Cults, da anni stanziati in Italia e organizzati in strutture gerarchicamente ordinate. Questi gruppi sono rimasti spesso coinvolti in violente contrapposizioni, nell'intento di espandere i rispettivi traffici illegali ed affermare la propria supremazia. Essi mantengono stretti contatti con omologhe formazioni presenti in Italia e in diversi Stati europei, oltre che con figure apicali stanziate in Nigeria, allo scopo di coordinarsi, per l'organizzazione interna e le strategie criminali da attuare nei rispettivi territori d'influenza. I sodalizi criminali nigeriani operano su buona parte del territorio nazionale, comprese le Regioni ove risulta forte il controllo della criminalità endogena, come ad esempio in Campania e Sicilia. Gli ambiti criminali di azione dei citati sodalizi sono il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e del lavoro irregolare. La tratta di esseri umani, finalizzata allo sfruttamento della prostituzione, è gestita da organizzazioni transnazionali con collegamenti in territorio africano ed europeo. Le ragazze nigeriane, reclutate in madrepatria con la promessa di un posto di lavoro in Italia, sono, di fatto, ridotte in schiavitù, anche mediante riti magico-tribali. Tali organizzazioni, inoltre, farebbero spesso ricorso alla figura della *maman* che, come emerso in diverse attività d'indagine, assume i ruoli di reclutatrice, organizzatrice, sfruttatrice, capo di unità operative, punto di raccordo fra i diversi strati dell'organizzazione, cassiera ed investitrice dei proventi delle attività illecite. II fenomeno è attentamente monitorato da parte delle Forze di polizia che, anche nel 2018, hanno concluso diverse operazioni di polizia giudiziaria. In particolare, a Palermo, Catania e in provincia di Napoli, tra marzo e maggio di quest'anno, sono stati arrestati diversi cittadini nigeriani (in totale 16) ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nonché di reati di tratta di essere umani nei confronti di giovani donne loro connazionali. Inoltre, nel luglio scorso, la squadra mobile della Polizia di Stato, coadiuvata da personale del reparto prevenzione crimine Umbria e Lazio, ha eseguito, a Perugia, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sette nigeriani, sottoponendo agli arresti domiciliari un altro nigeriano, ritenuti responsabili di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione aggravati dalla transnazionalità. Gli esiti dell'attività di contrasto al narcotraffico, esercitata dalle Forze di polizia, evidenziano che i nigeriani sono molto attivi anche in questo campo, in cui anche le donne svolgono diversi compiti. È accertato che la Nigeria costituisce uno snodo fondamentale nella rotta della cocaina dal Sud America verso l'Europa, e che gli apparati investigativi dei Paesi africani presentano alcune criticità. Tale situazione permette ai trafficanti di creare e gestire porti franchi in territorio nigeriano, anche grazie alla complicità di connazionali che vivono in vari Paesi del mondo e offrono idoneo supporto logistico. Per la fase più rischiosa del trasporto, i gruppi nigeriani preferiscono avvalersi di soggetti non strettamente legati all'organizzazione, utilizzando anche persone di altre nazionalità, impiegati come corrieri "ovulatori" per eludere i controlli doganali. Nel sistema del controllo delle piazze di spaccio, i nigeriani prediligono una gestione autonoma senza commistioni con altri gruppi attivi nel medesimo settore. Anche su questo versante l'attività di contrasto delle Forze di polizia è costante e particolarmente incisiva: nel giugno scorso infatti il servizio centrale operativo della Polizia di Stato, in collaborazione con la locale squadra mobile, ha eseguito a Perugia 28 arresti differiti nei confronti di un gruppo criminale composto, principalmente da nigeriani. L'operazione, denominata "Pusher 3-Piazza Pulita", ha disarticolato una piazza di spaccio attiva nel capoluogo umbro. Nel mese di luglio invece analoga operazione ha portato ad eseguire a Venezia un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 25 nigeriani, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, riciclaggio e decesso come conseguenza di altro delitto. Per quanto riguarda, poi, i delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, si è continuato a registrare l'interesse delle organizzazioni criminali di matrice nigeriana prevalentemente nei settori del traffico di valuta falsa, della clonazione ed indebito utilizzo di mezzi elettronici di pagamento nonché delle truffe per corrispondenza e per via telematica. Gli ingenti proventi conseguiti nelle attività illegali vengono successivamente inviati in madrepatria, anche attraverso reti di raccolta e trasferimento di denaro, tra le quali *money transfer* e *hawala* e, in misura minore, sono oggetto di riciclaggio, oppure vengono reinvestiti sul nostro territorio, principalmente in imprese che, per caratteristica e distribuzione, sono in grado di costituire punti di aggregazione per i connazionali e, quindi, utili strumenti di controllo per i traffici illeciti. A tal proposito, nell'agosto 2017, la Guardia di finanza ha condotto un'importante operazione tra le province di Milano, Bergamo, Brescia e Verona, denunciando, in stato di libertà, 9 nigeriani. L'indagine ha consentito di disarticolare un'organizzazione criminale, con solide ramificazioni in Nigeria, attiva nella raccolta di denaro proveniente dal traffico di stupefacenti e dallo sfruttamento della prostituzione, rimesso in madrepatria a mezzo di corrieri. Nel corso dell'operazione sono stati sequestrati circa 223.000 euro in contanti presso gli aeroporti di Fiumicino, Linate e Malpensa. Dal quadro delineato si evince come le Forze dell'ordine mantengano molto alto il livello di attenzione nei confronti del fenomeno criminale nigeriano che, come evidenziato, presenta peculiarità e caratteristiche di particolare pericolosità. La capacità di controllo di territori in cui già sono radicate forme di criminalità autoctone, la connotazione etnico-tribale, l'efferatezza dei metodi criminali utilizzati, impongono una strategia di contrasto basata su forme di collaborazione ed attività di indagini anche sul piano internazionale. In tale direzione, faccio presente che il Dipartimento della pubblica sicurezza ha intensificato la collaborazione investigativa con le autorità nigeriane per il controllo dei flussi immigratori e il contrasto del connesso fenomeno della tratta degli esseri umani. il Governo continuerà a riservare il massimo impegno nella strategia di contrasto di tali sodalizi criminali, come peraltro è evidenziato dai risultati registrati nel periodo giugno-luglio 2018, che hanno visto un incremento del dato relativo ai cittadini nigeriani denunciati ed arrestati per i reati di sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile cento), nonché per quelli connessi allo spaccio e al traffico di sostanze stupefacenti (più 1,34 il sottosegretario Molteni, ma non ci possiamo dichiarare soddisfatti. Il Sottosegretario ha fatto un lungo elenco dei crimini commessi dalla mafia nigeriana, ci ha confermato esiste una organizzazione mafiosa molto radicata e pericolosa, dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, al favoreggiamento della prostituzione, a crimini di ogni genere (non ha potuto citare l'omicidio di Pamela Mastropietro, ma sappiamo che anche in quel caso la mafia nigeriana ha avuto un ruolo) e ci ha elencato l'ottimo lavoro svolto dalle nostre Forze dell'ordine. La ringrazio, ma noi chiedevamo cosa intende fare il Governo per contrastare quello che è oggi un fenomeno molto pericoloso e la mafia emergente sul nostro territorio. Purtroppo continuiamo a notare una grave sottovalutazione del fenomeno della mafia nigeriana in Italia: lo abbiamo visto finora con i Governi precedenti, sui grandi *media* e da parte dei professionisti dell'antimafia pronti a denunciare ogni organizzazione criminale e a parlare di mafia in ogni contesto, in ogni parte del pianeta, tranne che di mafia nigeriana: rivolgiamo quindi da quest'Aula un appello a Roberto Saviano a dedicarsi anche alla mafia nigeriana, tra le varie cose che fa.

di persone che sbarcano sul territorio italiano e dire che ci sia una connessione tra l'immigrazione di massa illegale nigeriana e la mafia nigeriana rischia di creare un corto circuito in in chi sostiene l'immigrazione di massa in Italia. È questo il motivo per cui la sinistra, Saviano, tutti i professionisti dell'antimafia non hanno mai affrontato il problema della mafia della mafia nigeriana ed è il motivo per cui invece Fratelli d'Italia lo ha sempre fatto. Oggi però ci aspettavamo un cambio di passo che invece non vediamo. Si dice che tre indizi fanno una prova

e del mare*. Signor Presidente, onorevoli senatori, con riferimento alle questioni poste, sulla base degli elementi acquisiti, si fa presente in via preliminare che l'Impianto di trattamento e rifabbricazione elementi di combustibile (ITREC), che si trova all'interno del centro ricerche ENEA della Trisaia, è stato costruito fra il 1965 e il 1970 per ricerche sui processi di ritrattamento e rifabbricazione del combustibile uranio-torio. Nel 1987 le attività sono state interrotte e si è proseguito con il mantenimento in sicurezza degli impianti. Nel 2003 la Sogin ha assunto dall'ENEA la gestione dell'impianto con l'obiettivo di realizzare la bonifica ambientale e lo smantellamento del sito. Nel mese di febbraio 2017, a seguito di denuncia da parte di una ditta appaltatrice che lamentava anomalie e criticità nell'esecuzione dei lavori affidati dalla Sogin per l'esecuzione del piano di caratterizzazione del sito in questione, veniva iscritto dalla procura della Repubblica di Matera il procedimento penale n. 578 del 2017. Come riferito dalla prefettura, le indagini effettuate in merito hanno rilevato la condotta di scarico nel Mar Ionio di effluenti liquidi prodotti dall'impianto non risulterebbe autorizzata. Nel mese di aprile 2018 tutte le indagini sono state trasmesse per competenza alla procura della Repubblica di Potenza, che ha disposto il sequestro penale. Le condotte poste sotto sequestro sono due: una in area ENEA, in disuso, e una in capo a Sogin. Al riguardo, ISPRA ha precisato che il citato sequestro delle tre vasche del sistema di raccolta degli effluenti d'impianto e dell'associata condotta di scarico a mare riguarda la presenza di contaminanti chimici, riscontrata nell'acqua di falda, che viene prelevata dai pozzi di drenaggio dell'impianto ITREC e raccolta nelle vasche stesse. A seguito del sequestro, secondo quanto riferito dal Ministero dello sviluppo economico, la Sogin ha adottato tutte le azioni consentite volte alla progettazione e fornitura di un impianto di trattamento delle acque drenate dalla falda, che garantirà l'abbattimento delle sostanze inquinanti mediante processi chimico-fisici e ha inoltre realizzato un nuovo sistema di accumulo. In merito all'accertamento di contaminazione di tipo convenzionale nel sito relativo al superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione rilevato da Sogin durante il monitoraggio prescritto dall'AIA, l'ISPRA ha evidenziato che è in corso il procedimento di messa in sicurezza e bonifica, avviato dalla Sogin e dall'ENEA. La conferenza di servizi del 10 aprile 2018 ha approvato gli esiti dell'analisi di rischio presentata dalla Sogin stessa, che ha individuato come probabile fonte primaria di contaminazione una sorgente esterna al perimetro delle attività della suddetta società. A seguito di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, ISPRA si è espresso evidenziando la necessità, da parte del gestore del sito, di predisporre un trattamento delle acque emunte in grado di rimuovere la contaminazione riscontrata nelle acque drenate al di sotto dell'impianto ITREC. A ciò si aggiunga che l'ARPA Basilicata pone in atto un programma di monitoraggio ambientale indipendente. Detti programmi non evidenziano la presenza di anomalie radiometriche. L'ISPRA, nell'ambito dei suoi compiti di autorità di regolamentazione competente in ambito nucleare, ha svolto le proprie verifiche in relazione agli aspetti di sicurezza nucleare e di radioprotezione e si è espresso in merito all'efficacia del sistema di trattamento proposto dalla Sogin nel maggio 2018. A valle dell'istruttoria condotta, anche sulla base degli esiti dei sopralluoghi tecnici effettuati dai funzionari dell'istituto, si è ritenuto che l'impianto di trattamento non determina interferenze per la gestione in sicurezza e risulta rispondente ai requisiti di radioprotezione. In particolare, sono stati ritenuti idonei, ai fini dell'abbattimento delle sostanze inquinanti presenti nelle acque emunte dai pozzi di drenaggio nell'impianto ITREC, il trattamento chimico-fisico per la rimozione dei metalli pesanti e la filtrazione con carboni attivi per la rimozione dei composti organici e si è ritenuto condivisibile lo schema impiantistico proposto. Per quanto concerne, invece, il presunto sversamento nello Ionio di liquidi provenienti dall'impianto ITREC, il Ministero ha chiesto ad ISPRA di predisporre con la massima urgenza un idoneo piano di monitoraggio dell'area dell'area interessata dallo sversamento per valutare l'estensione e la gravità dell'inquinamento. Lo stesso Ministero, nel maggio 2018, ha richiesto ad ISPRA una verifica dello stato dei luoghi e una valutazione del danno ambientale in riferimento alla situazione che interessa la zona del citato impianto ITREC,

Alla stregua delle informazioni esposte, il Ministero dell'ambiente sta pertanto monitorando costantemente e in modo vigile la situazione di contaminazione e la minaccia di danno ambientale alle acque sotterranee. A tale riguardo, il Ministro ha recentemente rappresentato a tutti i soggetti interessati la necessità e l'urgenza che la Regione Basilicata proceda con gli accertamenti necessari all'individuazione delle fonti primarie di contaminazione, che l'ENEA provveda alla bonifica dell'ex impianto industriale Magnox, che Sogin continui, nei limiti fissati dall'autorità giudiziaria, nell'attività di *decommissioning* del proprio impianto e infine che il Sistema nazionale per la protezione ambientale disponga l'avvio di una campagna di monitoraggio delle acque marino-costiere, utilizzando appositi *biomarker*.

perché ha dato una risposta puntuale e attenta, che allo stato non può che soddisfarmi, soprattutto per la parte finale e dispositiva, laddove finalmente si fanno - come si suol dire - i nomi e i cognomi di chi deve fare cosa: cosa: l'ISPRA, che deve predisporre con la massima urgenza un piano di monitoraggio dell'area interessata dallo sversamento, per valutare l'estensione e la gravità dell'inquinamento; la Regione Basilicata, che - mi sento di dirlo anche in questa sede - non si è mai dimostrata, così come avrebbe dovuto, tanto sensibile alla tematica; e poi l'ENEA, la Sogin e l'SNPA.

ciò non dovesse succedere, serve una spinta che questo Ministero con le vostre persone può e sa dare, perché facciano finalmente il loro dovere. È mio compito, per adempiere al dovere morale che il mio ruolo mi impone, osservare in questa sede di cosa vive la Basilicata e, soprattutto, di cosa vive quella zona della Basilicata che è oggetto di questa contaminazione. Vive di turismo, soprattutto di turismo balneare, vive di agricoltura e vive anche di ambiente. Capirete tutti che che questi tre aspetti, che sono un importante volano per l'economia lucana (e non soltanto lucana, direi italiana), vanno a forte rischio laddove si dovesse parlare e verificare, come ahimè è accaduto in questo caso, di contaminazione ambientale.

L'agricoltura viene direttamente intaccata da questa attività, che non ha il controllo che merita; l'ambiente è un patrimonio che madre natura ci ha dato e che non può essere messo in discussione da nessun tipo di intenzione imprenditoriale, da chiunque sia stimolata e guidata, men che meno da queste attività, che rappresentano dei parcheggi che molte volte vengono attenzionati in aree come la nostra terra, cioè la Basilicata. Tra le varie le varie battaglie che a noi spetta combattere, c'è quella della disoccupazione, quella della tutela ambientale, quella delle infrastrutture, ma c'è anche una madre battaglia, quella della desertificazione, tanto ambientale quanto umana. Ambientale, perché noi siamo oggetto di perforazioni per fornire petrolio; ma anche umana, perché, ahimè, non essendoci infrastrutture, non essendoci occupazione e addirittura vedendosi minacciata da questi rischi, tanta gente va via e le famiglie non fanno più figli. Quindi, tramite

ai cimiteri nucleari di scorie (e non solo), perché la Basilicata ha già dato e non è più disposta a riceverne o a mantenerne di rischiosi così come potrebbe essere il caso che stiamo trattando. Un nuovo corso, signor Sottosegretario, che risponda al nome della verità e della giustizia.

là dove qualcuno ha sbagliato, deve pagare, perché queste ombre non possano e non debbano più addensarsi sulle nostre comunità *(Applausi

una nuova finestra"). L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento, alle quali risponderanno il Ministro della salute, il Ministro per la famiglia e le disabilità e il Ministro per il Sud.

la domanda è molto semplice, ma cade oggi che è il giorno dell'approvazione della Nota aggiuntiva al DEF, un primo passaggio che - mi auguro - sia finalmente di verità. La domanda è semplice: quale sarà il finanziamento del Sistema sanitario nazionale nel 2019 e nel triennio? La domanda nasce dalla necessità di fare chiarezza e di dare certezza ad un sistema che è in grandissima sofferenza. Tutti i dati ci parlano in modo univoco - siamo agli ultimi posti nel finanziamento UE-OCSE; sull'erogazione dei LEA vi sono profonde disuguaglianze, in tutto il sistema, anche nelle Regioni più efficienti, la qualità stenta; sul personale, come lei ben sa (e ho ascoltato anche le sue dichiarazioni), siamo all'emergenza; l'aspettativa di vita è alta ma la qualità diminuisce in modo significativo; cresce la spesa privata e siamo ormai a 40 miliardi

Gli investimenti in questi ultimi anni sono al palo. Abbiamo strutture che non solo non sono antisismiche,

Serve certamente un progetto di rilancio del sistema sanitario, rilanciando l'ispirazione originaria che quaranta anni fa produsse quella che credo sia la riforma più importante della storia della Repubblica italiana.

l'investimento di questo Governo per la sanità? Signor Presidente, inizio con una breve riflessione: ritengo che le ragioni dell'andamento decrescente del rapporto tra spesa sanitaria e PIL sono da ricercare nell'andamento dello stesso PIL, previsto in sensibile aumento rispetto a quanto avvenuto negli anni scorsi, in termini sia tendenziali sia programmatici, con un incremento per gli anni 2018-2021 anche in misura superiore rispetto ai valori già scontati nel DEF relativo al 2017. Quanto all'incremento del livello di finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato, l'incremento di quest'ultimo risulta collegato al recente andamento della spesa sanitaria. A tal proposito, ritengo opportuno ricordare che, proprio a fronte delle voci di costo che caratterizzeranno ancora nell'immediato futuro l'andamento della spesa sanitaria (acquisto di farmaci ospedalieri e, in particolare, spesa per farmaci innovativi - antiepatite C - e per farmaci innovativi oncologici) nello stato di previsione del Ministero della salute sono stati istituiti due fondi per il concorso al rimborso alle Regioni della spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e per l'acquisto dei farmaci innovativi oncologici. Come è noto, le risorse statali non esauriscono l'intera disponibilità di fondi delle Regioni chiamate ad erogare assistenza e servizi sanitari: al finanziamento statale, infatti, vanno aggiunti i ricavi derivanti dalla compartecipazione del cittadino per fruire sia di talune prestazioni di assistenza specialistica, sia di assistenza farmaceutica, nonché il gettito fiscale di cui beneficiano le Regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, cioè la massimizzazione delle aliquote IRPEF e IRAP. È possibile quindi affermare che il descritto il rapporto tra finanziamento e spesa del Servizio sanitario nazionale fornisce adeguate garanzie in merito alla sostenibilità del sistema. Peraltro segnalo che per l'anno 2019 il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario *standard* a cui concorre lo Stato sarà incrementato almeno di un miliardo di euro rispetto alla disponibilità del 2018. Tuttavia, nella consapevolezza che i livelli delle prestazioni sanitarie sono determinati dalla funzionalità e dalla crescita del sistema sanitario attraverso nuovi interventi e nuovi progetti, adeguati alle caratteristiche del nostro sin dal mio insediamento al Ministero della salute ho intrapreso iniziative finalizzate ad individuare le misure più urgenti da adottare nell'attuale quadro di riferimento. In particolare, per quanto riguarda il personale della sanità, devo rammentare che la legge di stabilità per il 2017 aveva previsto, nazionale (FSN) il vincolo delle risorse necessarie a garantire il rinnovo dei contratti riguardanti il personale dipendente e convenzionato col Servizio sanitario nazionale, senza tuttavia prevedere a tale scopo un incremento dello stesso Fondo. Quindi stiamo lavorando su questo. Pertanto, in sede di rinnovo dei contratti collettivi nazionali è emersa l'insufficienza delle risorse per garantire i benefici contrattuali. Ecco perché rinnovo anche in questa sede il mio impegno e verificare, nell'ambito della prossima manovra finanziaria, la possibilità di individuare le risorse necessarie sia al riconoscimento dei benefici contrattuali, sia ai fabbisogni assunzionali, anche in considerazione della fuga dei professionisti dal Servizio sanitario nazionale, che si è registrata negli ultimi anni, nella consapevolezza che avviando un'efficace politica per il personale potrà essere incrementata e potenziata l'attrattività dell'intero sistema sanitario nazionale.

Ministro, prendo atto delle sue parole in relazione all'impegno per quanto riguarda il contratto e le spese del personale. Tuttavia non posso che esprimere la mia profonda insoddisfazione sulla prima parte del suo ragionamento che

di tagli e di un definanziamento per il funzionamento del sistema sanitario tra il 2015 e 2018 di 12 miliardi; cifra che, se la si prende dal 2010 al 2018 (e non solo dal 2015 al 2018) arriva a 40 miliardi. La spesa sanitaria italiana, a seconda che la si valuti a parità di potere d'acquisto o meno, è sotto la media dell'Europa occidentale tra il 25 e il 31,2 C'è un definanziamento strutturale della sanità che, anche con il miliardo in più - come le ho già detto - e con un riconoscimento delle spese contrattuali, porterà il sistema in una situazione di grave difficoltà. E visto che nel contratto ci sta scritto che volete tutelare il sistema sanitario nazionale, veramente lo volete tutelare, occorre un investimento strategico, triennale. Poi la lotta agli sprechi e quegli sprechi e quei risparmi vanno reinvestiti in sanità.

si è stabilito che si può presentare una dichiarazione sostitutiva della documentazione originale per le vaccinazioni entro il 10 marzo 2019, rinviando quindi questo obbligo. Per i bambini immunodepressi si vede leso il diritto all'istruzione, si va a indebolire la parte più fragile della popolazione per favorire i figli dei genitori no vax per motivi puramente elettorali. In uno Stato di diritto si dovrebbe garantire l'istruzione a tutti.

vaccini, all'articolo 5 si dice che i piani straordinari d'intervento saranno solo in presenza di emergenze sanitarie o di «significativi scostamenti dagli obiettivi». Vorremmo capire cosa si intende per «significativi scostamenti» e su quali evidenze scientifiche

noi le poniamo alcune domande in modo molto chiaro e la pregherei, se possibile, di risponderci in modo altrettanto chiaro, possibilmente non leggendoci il compitino scritto o comunque leggendolo più lentamente, visto che in quest'Aula si si fa la diretta anche per far capire ai cittadini che cosa stiamo dicendo e ho difficoltà a credere che i cittadini abbiano capito la risposta alle domande precedenti. Quante volte avete cambiato idea? Che posizione avete su questo tema? I cittadini hanno il diritto di saperlo in modo chiaro; anche noi. Cosa significa obbligo flessibile? Cosa si vuol fare per ripristinare l'evidenza scientifica e tutelare la sicurezza collettiva? Che iniziative avete intenzione di intraprendere per consentire, fino al 10 marzo, il diritto all'istruzione dei bambini immunodepressi? E dopo il 10 marzo coloro che non avranno presentato la dichiarazione sostitutiva vedranno precluso l'accesso alle scuole dell'infanzia? Noi vogliamo sapere cosa succederà prima del 10 marzo, cosa succederà dopo, che cosa si intende per obbligo flessibile, qual è la vostra posizione sul tema delle vaccinazioni, perché ancora, in tre mesi, non l'abbiamo capito e abbiamo sentito tutto e il contrario di tutto.

ringrazio gli onorevoli interroganti in quanto consentono di precisare il mio pensiero in tema di obbligo vaccinale. Sono convinta che l'obbligo, pur necessario, debba comunque tenere conto della situazione epidemiologica che si registra in un dato contesto territoriale o in determinate comunità o in relazione a categorie di individui. L'obbligo è uno strumento di politica vaccinale ed è questo lo schema che seguono anche Paesi come la Spagna e la Germania. Obbligare alle vaccinazioni può essere necessario, dunque, ma non è sufficiente ai fini di prevenzione; lo dimostra l'epidemia di morbillo in corso nel nostro Paese e l'aumento delle coperture, che l'obbligo ha prodotto nelle generazioni di nuovi nati, non ha interrotto la diffusione della malattia. Infatti, l'eliminazione del morbillo richiede l'attuazione di un complesso di interventi, descritti in un piano già disponibile e che è stato tuttavia colpevolmente dimenticato dal 2011, oltre che non finanziato. Per interrompere l'epidemia occorre, per esempio, promuovere la vaccinazione fra gli operatori sanitari, per garantire le occasioni di contatto con i servizi sanitari, e occorre potenziare molto la comunicazione sociale. Per questo intendo aggiornare rapidamente il piano morbillo - cosa che avrebbe dovuto fare il precedente Governo e non ha fatto - e proporre al Governo e alle Regioni di assumersi impegni concreti, trasformando le raccomandazioni del piano in azioni finalizzate e verificabili. In questo senso, è apprezzabile l'iniziativa del disegno di legge parlamentare di maggioranza, che mira a completare la normativa vigente. Auspico che siano previste iniziative concrete, come potenziare i servizi vaccinali, così come ci chiede l'Organizzazione mondiale della sanità; rendere operativa l'anagrafe nazionale vaccinale, che manca ancora in questo Paese, colpevolmente; monitorare le coperture agli eventi avversi e finanziare adeguatamente la spesa. Tra i tanti strumenti non dovrebbe mancare anche quello dell'obbligo, naturalmente, ove la situazione epidemiologica ne indichi i presupposti. Saranno gli organi istituzionali dello Stato e delle Regioni a stabilire per quali vaccini e per quali popolazioni varrà l'obbligo. Anche per i bambini immunodepressi, la cui tutela mi sta particolarmente a cuore, è sbagliato puntare solo all'obbligatorietà e chi lo fa credo che operi in modo strumentale, perché al momento, per le fasce di età scolare, permane esattamente il regime previsto dal decreto-legge Lorenzin e, poi, perché la vaccinazione dei compagni di classe non basta a proteggere contro tutti i rischi cui sono purtroppo esposti questi bimbi. Come ci ha ricordato il Centro nazionale dei trapianti, la loro protezione richiede progetti personalizzati, che tengano conto di tutti i rischi ambientali e non solo di quelli scolastici, delle loro difese residue e delle loro capacità di controllare le relazioni, affinché crescendo imparino a proteggersi e a evitare rischi. Anche l'ultima domanda è strumentale, atteso che con il decreto-legge milleproroghe non si è fatto altro che prorogare un regime già previsto per lo scorso anno scolastico dal decreto-legge Lorenzin. Pertanto, a legislazione vigente, in maniera molto semplice, dopo il 10 marzo 2019 avranno accesso alle scuole dell'infanzia e ai servizi educativi per l'infanzia i minori i cui genitori daranno prova di quanto già dichiarato mediante la presentazione del libretto vaccinale o di altra documentazione idonea.

inventato l'obbligo intelligente, l'obbligo federale, l'obbligo flessibile, l'obbligo alternato, l'obbligo morbillo sì, esavalente no. Grazie a voi l'obbligo scolastico è diventato l'obbligo di stare a casa per i bambini immunodepressi 10.000 bimbi che avrebbero il diritto di andare a scuola senza rischiare la vita non potranno farlo a causa dell'ignoranza e dell'egoismo di chi non vaccina e di un Governo che gli strizza l'occhio. Non dovrebbe essere fatta alcuna mediazione con i no vax, nessuna sfumatura: così come chi fuma non può entrare al cinema, chi non è vaccinato non può entrare in classe. Punto e basta. Avete cavalcato e promosso le bufale contro i vaccini, con il vostro uso fasullo e malato dei *social*. Siamo arrivati ad una copertura sul morbillo sotto Zambia e Sudan, ci avete costretti al decreto Lorenzin, un provvedimento duro ma necessario, e ora fate gli splendidi liberali. Avete giocato con la salute la salute dei bambini per prendere i voti dei no vax*.* Libertà non è potere di danneggiare gli altri in nome dell'egoismo e della superstizione, la libertà è un'altra cosa. Avete scambiato la libertà per la tirannia dei no vax. Uno Stato di diritto non è quello in cui ognuno fa come gli pare così come avete fatto. La libertà individuale trova un limite in quella altrui e lo Stato deve garantire questo equilibrio senza cedimenti. Come per l'ILVA, per il ponte di Genova e per tutto quello che avete detto e non fatto, il Paese è vittima della vostra lenta, faticosa, pericolosa, comica inversione ad ma non fate ridere più nessuno. Ve ne siete fregati del clima di incertezza e del caos causato alle famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti scolastici e ai medici,

Ricordo soltanto che le interrogazioni non sono uno strumento dell'opposizione, ma espressione di istanze dei cittadini che chiedono risposte soprattutto per i pazienti. Detto questo, Detto questo, l'autocertificazione voluta dal Governo sulle vaccinazioni obbligatorie fino al 10 marzo 2019 reca una serie di contraddizioni e non è chiaro quali saranno gli effetti in caso di inadempimento. Forza Italia, che da sempre ha fatto una battaglia di civiltà su questo tema, considera che sia stato fatto un passo indietro rispetto alla valorizzazione dell'obbligo vaccinale, mentre il Governo ha introdotto la proroga solo per mantenere promesse elettorali, senza tenere conto del parere della scienza, dei problemi che avranno i dirigenti scolastici delle ripercussioni sui bambini e sulle loro famiglie e sulla salute pubblica. Le vaccinazioni sono un pilastro per la sanità, perché consentono di prevenire malattie infettive gravi che possono portare complicanze e la morte. Il rischio di reintroduzione di malattie è maggiormente presente per l'Italia, aperta al Mediterraneo e al centro di flussi migratori privi di controllo sanitario. Se le coperture vaccinali continueranno a scendere, sarà inevitabile il ritorno di alcune malattie anche nel nostro Paese. Per la inadeguata copertura vaccinale, sappiamo che nel 2017 ci sono stati 5.000 casi di morbillo, ma Ministro, lei è un medico, non può pretendere che in un anno di obbligo vaccinale la malattia scompaia. I vaccini servono a questo, ci vuole del tempo e le emergenze, come detto nelle supposto disegno di legge, non si sa bene a che punto devono iniziare. Ricordo anche che lo Stato polio *free* in Europa non c'è più, basta vedere le dichiarazioni del 2017 del commissario europeo per i casi in Pakistan, Afghanistan e Albania. Questa situazione mette a rischio i bambini immunodepressi e tutti i trapiantati; certamente non li mette a rischio di altro, ma almeno elimina parecchi rischi.

In ogni caso la domanda riguarda il vaccino esavalente, che lei ha solo raccomandato. Questa affermazione contravviene all'indicazione del mondo scientifico e io ritengo molto grave e inaudito che lo dica un Ministro e soprattutto un medico. Le chiedo perciò di chiarire in maniera definitiva come intende procedere per le malattie comprese nella vaccinazione esavalente: poliomelite, tetano, pertosse, epatite B, haemophilus (che comporta anche la meningite) e la difterite, che al giorno d'oggi sono ancora malattie mortali, come testimoniano i casi degli anni scorsi in Francia, Spagna

Con particolare riguardo all'autocertificazione e ai rischi potenziali ad essa correlati, mi preme sottolineare che con l'emendamento al decreto-legge milleproroghe è stato semplicemente esteso all'anno scolastico in corso il regime transitorio già previsto dal decreto-legge Lorenzin, lo ripeto: il regime transitorio

l'azienda sanitaria territorialmente competente spesso non dispone delle informazioni aggiornate sullo stato vaccinale di tutti i minori. In definitiva, l'autocertificazione si spiegava e si spiega in considerazione della assenza dell'anagrafe nazionale vaccini, il cui decreto istitutivo è stato da questo Ministero appena

nel senso che metterà a disposizione tutte le informazioni necessarie sia per poter verificare tempestivamente la reale effettuazione delle vaccinazioni, sia per compiere un'istantanea valutazione del livello di copertura su tutti i territori, in modo da avviare interventi mirati al raggiungimento degli obiettivi immunologici. Quanto alle false autocertificazioni, ribadisco quanto detto di nuovo in altre occasioni. Semplificare, agevolando le modalità di autocertificazione non significa sostenere chi intende dichiarare il falso;

con l'evoluzione normativa che da anni ormai privilegia il principio di fiducia in luogo di quello del controllo preventivo. Inoltre, il Ministero della salute ha già ulteriormente rafforzato le verifiche relative alla veridicità delle dichiarazioni. Peraltro, da un lato, i dati a disposizione dimostrano che su oltre 55.700 antisofisticazione e sanità (NAS) di recente, solo lo 0,09 per cento del totale delle autocertificazioni ma anche delle certificazioni non corrisponde al vero; dall'altro, proprio come si evince da questi controlli, sulle dichiarazioni dei genitori relative alle situazioni vaccinali dei propri figli minori risultano non veritieri indifferentemente sia i certificati che le dichiarazioni sostitutive. Per questo si ha modo di ritenere che purtroppo il problema dell'onestà non riguarda soltanto le autocertificazioni. Concludendo, dalla proroga della possibilità di autocertificare e dall'implementazione dell'anagrafe nazionale, il Governo si attende di migliorare il rapporto scuola-famiglia, agevolando la frequenza a tutte le scuole e agli asili nido, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa e - mi preme ribadirlo - senza pregiudizio alcuno per l'interesse pubblico alla tutela della salute.

immagino che abbia certamente fatto la tipizzazione degli anticorpi per la rosolia, dal momento che è una di quelle malattie del complesso TORCH che provoca numerose malformazioni nei bambini. Per quanto riguarda la domanda sul vaccino esavalente, a pagina 11 dell'ordine del giorno

pochi mesi fa a Bergamo. Signor Ministro, abbia il coraggio di cambiare ancora una volta idea, gliene saremmo tutti grati, anche i figli dei no vax.

Abbiamo condiviso e suggerito molte soluzioni ai problemi che la famiglia deve affrontare e da cui è minacciata. La famiglia si confronta ogni giorno con la riduzione della natalità, l'invecchiamento delle persone, la mancanza di strutture a supporto e la perdita del potere d'acquisto

lo schieramento di centrodestra ha condiviso c'era l'istituzione di un reddito dedicato alle famiglie con figli numerosi, l'introduzione del quoziente familiare, la previsione di agevolazioni fiscali per i prodotti per la prima infanzia, il rafforzamento del congedo parentale,

se queste proposte saranno accolte dal Governo e troveranno ospitalità nei prossimi provvedimenti.

ringrazio l'interrogante per avermi dato l'opportunità di ribadire il valore fondamentale della famiglia e della natalità, sancito dalla Costituzione e che ha riflessi positivi sia dal punto di vista economico, che da quello della riduzione del debito pubblico. Mi piace sottolinearlo in particolare in queste ore di definizione delle linee di bilancio della Nota di aggiornamento al DEF. Negli ultimi anni le famiglie italiane sono state purtroppo severamente colpite dalla crisi economica e ciò ha contribuito ad acuire il crollo demografico, che, abbinato all'invecchiamento della popolazione, costituisce forse il principale problema strutturale del Paese, anche nella prospettiva degli equilibri di bilancio di medio e lungo termine. I dati dell'ultimo *aging report* della Commissione europea prevedono per l'Italia un tasso di fertilità pari a 1,42 figli per donna nel 2030, ben al di sotto della soglia di mantenimento. Sono quindi ben consapevole della necessità indifferibile di invertire la dinamica demografica avversa, considerando a tal fine le risorse spese in favore della famiglia e del sostegno alla natalità come veri e propri investimenti nel capitale sociale. In questa prospettiva e in vista della definizione della legge di bilancio, ho presentato un pacchetto di proposte al Ministero dell'economia per il rilancio della natalità e il sostegno alla genitorialità, che vertono sia sul versante fiscale, sia su quello dei servizi e delle prestazioni sociali. Apprendo con favore che molte iniziative proposte dall'interrogante corrispondono a quelle che stiamo già portando avanti: mi riferisco a misure come la definizione di un sistema fiscale a misura di famiglia; la possibilità di lasciare maggior reddito nelle disponibilità dei genitori, soprattutto di quelli con diversi figli a carico; il rafforzamento dell'istituto del congedo parentale; l'attenzione ai *caregiver;* l'incentivazione degli investimenti nel *welfare* aziendale e familiare; il rafforzamento della rete dei servizi a sostegno della famiglia e le agevolazioni per la loro più ampia fruizione, con particolare riferimento agli asili nido e alle strutture, anche private, per l'assistenza all'infanzia, senza considerare le politiche antidroga, che sicuramente attengono anche alla tutela delle famiglie e della genitorialità. Con riferimento all'istituzione di un reddito di infanzia richiamato dall'interrogante, ritengo che sia indispensabile definire un sistema di incentivi anche economici alla natalità e per la prima infanzia di carattere strutturale, da calibrare in modo selettivo e in un congruo arco temporale. Ho proposto infine di introdurre specifiche forme di tutela in favore dei soggetti che, in conseguenza di crisi familiari, versano sempre più spesso in condizioni di vulnerabilità socio-economica, nonché di potenziare il fondo per le politiche della famiglia, rivisitando anche le finalità cui lo stesso è destinato. Mi auguro che tutti i membri del Governo abbiano la mia stessa sensibilità rispetto ai temi della famiglia e della natalità e devo dire che ho riscontrato in diversi Ministri una notevole sensibilità nei loro riguardi, senza i quali, al di là di tutte le proposte che stanno emergendo in questi giorni nel dibattito sulla manovra finanziaria, io credo sinceramente che non sarà possibile far ripartire veramente il Paese.

Ministro, lei ha usato nelle sue dichiarazioni pubbliche e programmatiche anche in Commissione qui al Senato - gliene do atto - espressioni piuttosto forti riguardo alla sua volontà di dare un segnale di cambiamento. del fatto che bisogna investire maggiormente per i giovani, per la casa e per l'accesso al credito immobiliare; ha parlato della necessità di dare risposte ai milioni di famiglie che hanno una persona disabile e di tante altre cose che purtroppo non ho il tempo di ricordare. Il nostro compito, il compito del nostro Gruppo Fratelli d'Italia, che ribadiamo anche in questa occasione, è vigilare affinché le sue non rimangono soltanto Noi non pretendiamo tutto e subito, ma neanche poco o niente. Il nostro compito è vigilare affinché l'istituzione del Ministero per la famiglia e per la disabilità, che anche noi abbiamo voluto e per il quale abbiamo dato un voto favorevole, non si traduca

iniziamo a parlare di politica di coesione, ma cerchiamo anche di avere una prospettiva futura. Signor Ministro, lei sa benissimo che la Commissione europea, in data 29 maggio 2018, ha presentato la nuova proposta di regolamento comunitario n. 375 che riguarda il nuovo piano di sviluppo regionale e politica di coesione per gli anni 2021-2027. Esso individua al suo interno cinque obiettivi da perseguire. Il primo di questi è un'Europa più intelligente mediante l'innovazione, la digitalizzazione, la trasformazione economica e il sostegno alle piccole imprese e io sottolineo le piccole imprese perché l'Italia - lo sappiamo - è fondata su questo tipo di

e priva di emissioni di carbonio noi del MoVimento 5 Stelle da anni ci battiamo sulla de carbonizzazione; é quindi un ulteriore *assist* che non dobbiamo grazie all'attuazione dell'Accordo di Parigi e agli investimenti nella transizione energetica pulita, nelle energie rinnovabili e nella lotta contro i cambiamenti climatici. Al punto 3 abbiamo un'Europa più connessa dotata di reti di trasporto e digitali strategiche. In riferimento alle reti, vorrei sottolineare che a noi interessano le reti che riescano a colmare quel grande *gap* che registriamo tra le Regioni del Sud Italia

un'Europa più sociale che raggiunga risultati concreti riguardo al pilastro europeo dei diritti sociali. Al punto 5 c'è un'Europa più vicina ai cittadini che sostenga strategie di sviluppo gestito a livello locale e uno sviluppo urbano sostenibile in tutta l'Unione europea.

verde. Vista la storica difficoltà italiana nella gestione dei fondi comunitari, che ha ripetutamente portato alla parziale restituzione degli stessi, data l'incapacità dell'amministrazione regionale e centrale nell'assorbire e investire la totalità dei fondi a disposizione del nostro Paese; considerato l'impegno dimostrato dal Governo e in particolare dal Ministero da lei rappresentato, per una più corretta ed efficiente gestione dei fondi relativi al piano 2014-2020 quali azioni, nuove procedure di controllo e supporto e quali attività il Governo intende mettere in campo per una gestione il Governo intenda mettere in campo per una gestione corretta, efficiente ed efficace dei fondi destinati al nostro Paese, in modo da impedire sprechi ed assicurare l'utilizzo degli stessi per progetti realmente in grado di favorire la convergenza

ovvero diverse centinaia di milioni rischiavano di essere persi e, quindi, si rischiava di perdere diversi rimborsi. a favore del pubblico che ci ascolta da casa e quindi dei cittadini, che le risorse dei fondi strutturali europei non sono altro che risorse provenienti dallo Stato, e quindi dall'Italia e dai contribuenti italiani, che vengono in maniera

dalla scadenza entro la quale si deve rendicontare il primo *target* per ottenere rimborsi. La politica di coesione in realtà è sempre stata trattata con molta distrazione e non, purtroppo,

che - ahimè - ancora restano indietro. Con questo voglio dire che negli ultimi anni si è sostituita la spesa ordinaria per gli investimenti con la spesa di coesione, quella che doveva far recuperare il *gap*.

di tutti i componenti della maggioranza di Governo, avremo un'arma in più da mettere in campo, insieme ai Ministri di riferimento, per dare veramente una spinta

«Abolire la miseria»: così si intitolava lo splendido libro che l'economista Ernesto Rossi, autore, con Altiero Spinelli e Eugenio Colorni, de «Il Manifesto di Ventotene», scrisse in carcere nel 1942, e pubblicò nel 1946: «Bisogna unire tutte le nostre forze per combattere la miseria per le stesse ragioni per le quali è stato necessario in passato combattere il vaiolo e la peste: perché non ne resti infetto tutto il corpo sociale». La sfida oggi è identica, e sono le pubbliche istituzioni nazionali ed europee a doversi assumere questo grave compito. purtroppo, persino la sinistra ha dimenticato i poveri e preferisce prendere in giro chi, invece, ha quell'intento. Si fa riferimento naturalmente alla miseria materiale, che rende impossibile la vita di chi è costretto a una triste condizione, ma si fa riferimento anche alla miseria dell'animo dell'uomo, dell'indifferenza rispetto alle tragedie degli altri. Risalendo indietro nel tempo, il commediografo romano Terenzio faceva parlare così uno dei suoi personaggi nella commedia «Il punitore di se stesso», quando questi veniva invitato a non occuparsi che dei fatti suoi: «*Homo sum, humani nihil a me alienum puto*», nulla che sia umano mi è estraneo. Anche più recentemente, oggi, nel film del regista romano Luigi Magni, «In nome del popolo sovrano», Nino Manfredi interpreta il carrettiere Ciceruacchio, uno dei protagonisti della Repubblica romana del 1849. del 1849. Il personaggio risponde all'arrogante inquisitore, che gli domanda perché lui, misero carrettiere, si è impicciato di quella storia tanto più grande di lui: «Vede, eccellenza, io so' carrettiere, ma a tempo perso so' omo. E l'omo se impiccia! ». Così rispondeva. Questo è il modo di rispondere alla miseria umana, a quel cinismo che fa perdere la speranza e l'attenzione per i poveri e i fragili e si incarna anche nelle tristi ironie